Comunico che in data 31 ottobre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

vi prego di farlo perché l'argomento con cui apriamo i lavori credo meriti condivisione. Care senatrici e cari senatori, sapete - come me e meglio di me - che nella notte di giovedì 2 novembre una forte ondata di maltempo si è abbattuta

Il Consiglio dei ministri ha stabilito di destinare le prime risorse. Ma quel che più conta è che noi dobbiamo la la nostra gratitudine e il nostro plauso agli oltre 3.000 operatori tra Protezione civile, volontari, Vigili del fuoco, Forze di polizia e Forze armate, provenienti da diverse Regioni d'Italia, impegnati senza sosta in un lavoro encomiabile. Sappiamo benissimo che le forze della natura sono difficilmente del tutto imbrigliabili. Sappiamo che c'è un dibattito in corso sulle modifiche permanenti o temporanee del clima. Quello che però è sicuro, almeno per quanto attiene a chi non vuole in questa sede entrare in tale dibattito, è che occorre impegnare tutte le Istituzioni, da quelle centrali a quelle locali, affinché si realizzino opere di prevenzione strutturale e non strutturale

sono i *boy scout*, sono le case del popolo, sono le parrocchie. Uniamo però due considerazioni ulteriori a questo, signor Presidente, che affidiamo a lei e, per suo tramite, alla Sottosegretaria e al Governo: questa tragedia ha colpito il cuore della Toscana, la piana che va da Campi Bisenzio a Quarrata e che ha l'epicentro in quello straordinario comune che è il Comune di Prato. Prato è molto di più che un Comune: Prato è un esempio; Prato ha insegnato al mondo cosa vuol dire lavorare duro; Prato è un esempio di civiltà e di tenacia incredibile. La gente di Prato è tosta.

vogliono incentivi per gli acquisti delle aziende tessili che sono state distrutte. Signor Presidente, la prego di aiutarci a ricordare al Governo, che è andato per bocca del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri a promettere 300 milioni di euro - speriamo che siano veri che quello che chiede la gente di Prato è poter ripartire subito e ripartire con il lavoro. Se c'è infatti un'esperienza che da Prato è venuta a tutto il Paese - non importano i libri di Edoardo Nesi per ricordarlo - è che noi siamo persone che sanno che cosa vuol dire far fatica e ripartire. Contemporaneamente però, signor Presidente, mi lasci dire in conclusione che non ci può essere da parte di tutti noi, senza alcuna polemica, e da parte del Governo per il sovrappiù di responsabilità che gli compete, un ulteriore un ulteriore ritardo nell'unità di missione sul dissesto idrogeologico. Signor Presidente, nel momento in cui noi piangiamo le vittime di Prato e di tutta la Toscana, ci sono due opere pubbliche che hanno salvato due tra le principali città d'arte di questo Paese. Il Mose ha salvato Venezia, alla faccia di quelli che si lamentavano. Se non ci fosse stato il Mose, Venezia sarebbe finita sott'acqua il 2 novembre.

Anche a Prato alcune realtà - penso a Poggio a Caiano e Galciana - hanno subito meno danni di altri Comuni perché sono state fatte della casse di espansione e laminazione. siccome le opere pubbliche quando si fanno e stanno anche nel PNRR salvano vite, la prego ci aiuti a ricordar al Governo che l'unità di missione sul dissesto idrogeologico è una cosa da fare e non da rinviare, altrimenti le nostre sono solo lacrime di coccodrillo. La ringrazio. È presente un rappresentante del Governo, ma sarà mia cura sollecitare l'attenzione al suo intervento.

e naturalmente anche al ringraziamento per tutti quelli che in queste ore hanno dato una mano in tutte le maniere possibili per cercare di risolvere o comunque di contribuire a risolvere la drammatica situazione con la quale ancora una volta ci si è confrontati.

abbiamo proseguito con le Marche, poi c'è stata Casamicciola e ora c'è la Toscana. È la quarta volta nel giro di pochi mesi. Presidente, è del tutto evidente che siamo in presenza di un'anomalia rispetto al passato. C'è sempre stata la furia della natura. Ma il fatto che questa furia della natura si sia determinata in quattro volte, con così tante vittime, nel corso di così poco tempo,

con la quale bisogna fare i conti. Anche io penso che la politica non può semplicemente commemorare. Oggi è giusto che commemoriamo, ci stringiamo attorno alle vittime e osserviamo il nostro minuto di silenzio. Noi siamo però anche il Parlamento nazionale quindi, oltre a osservare il minuto di silenzio, mi piacerebbe molto per esempio fare una bella legge sul clima - come c'è in tanti Paesi d'Europa e non c'è invece in Italia - o una legge contro il consumo del suolo, come c'è in tanti Paesi d'Europa e non in Italia. Altrimenti, Presidente, le nostre rischiano di essere purtroppo lacrime di coccodrillo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretaria, ancora una volta la Toscana, la mia terra, è stata ferita a morte dalla violenza di piogge straordinarie che hanno colpite le province di Firenze, Prato e Pisa, il pomeriggio di giovedì 2 novembre. L'ultima vittima, l'ottava, poco fa: Antonio Tumolo, 84 anni, di Prato. di Prato. Giovanna Innocenti, 83 anni, di Livorno; Alfio Ciolini, 85 anni, di Montemurlo; Teresa Perrone, 65 anni, di Lamporecchio; Antonino Madonia, 70 anni, di Lamporecchio; Teresa Pecorelli, 84 anni, di Montemurlo; Gianni Pasquini, 69 anni, di Campi Bisenzio; Tindaro D'Amico, 73 anni, di Prato, hanno perso la vita nel tentativo di mettersi in salvo dalla furia di questa ennesima alluvione. Ai loro familiari esprimo la mia sentita vicinanza; a loro va il cordoglio mio e quello del Gruppo Forza Italia. Ancora una volta la nostra Regione - come nel 1966 e come altre volte negli ultimi decenni - è stata sconvolta e violata da quegli stessi elementi naturali che caratterizzano da sempre il suo straordinario paesaggio e la sua storia economica. Oggi non è il giorno delle polemiche: oggi è il giorno del dolore. Certamente, il dissesto idrogeologico del nostro Paese è un tema sempre più drammatico e urgente, e deve essere affrontato su scala nazionale. L'alluvione ha allontanato dalle proprie case 1.200 persone e causato danni stimati per 300 milioni di euro a una delle zone più produttive della Toscana. Anche adesso, in queste ore, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, che ringraziamo per il loro impegno senza sosta, stanno lavorando fianco a fianco ai tanti volontari e cittadini che non si sono persi d'animo, che in una corsa contro il tempo stanno collaborando per mettere in sicurezza i più fragili e che vogliono vedere presto le loro case, le loro città, le loro aziende tornare a una difficile normalità. Il nostro Governo è vicino alle popolazioni colpite. Ieri, a Prato, il vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha voluto dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese del territorio, mettendo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano; 200 milioni di prestiti agevolati e la sospensione fino al 30 giugno 2024 dei pagamenti sui finanziamenti. Il presidente Giorgia Meloni e tutto il Governo seguiranno giorno per giorno gli sviluppi di questo evento drammatico per elaborare strategie di intervento strutturale ed economico, ascoltando gli amministratori delle aree alluvionate e il governatore della Toscana Giani, nominato commissario straordinario. Alla mia Regione, alla nostra gente di Toscana, volitiva e ostinata, riservata ma caparbia, vanno il nostro abbraccio e da quest'Aula un messaggio: considerateci dalla vostra parte, noi ci siamo, ce la faremo, ce la farete.

eccoci qui, ci risiamo. Mi unisco al cordoglio per le vittime, all'apprezzamento e alla stima per l'intervento della Protezione civile e di tutti i volontari. Ma - ahimè - non posso che rilevare, come qualcun altro ha già fatto, che questo appuntamento sta diventando ricorrente. rischia di essere una sorta di lacrime del coccodrillo. Se non ci si decide a muoversi prima che il danno si produca e non solo dopo, non riusciremo a venirne a capo.

sono cambiati e quindi, piove tanto in pochissimo tempo e il suolo non riesce ad assorbire, anche perché è cementificato. Il rapporto di assorbimento tra un suolo cementificato e uno naturale è di uno a sei, nel senso che quello naturale assorbe sei volte di più l'acqua che scende. Quindi, con il suolo cementificato, l'acqua acquista una forza, una velocità e una violenza tale da procurare immensi danni. La piana toscana da Pistoia a Firenze è una naturale vasca di laminazione per i corsi d'acqua che scendono dell'Appennino, ma - ahimè - è stata cementificata in gran parte. Oltretutto, la Toscana è una terra di frane

nuovo hanno edificato, ma nessuno pare preoccuparsene. Si indossal'uniforme della Protezione civile, mentre i Presidenti delle Regioni e i sindaci dovrebbero indossare l'uniforme della prevenzione civile prima della prossima alluvione. Occorre fermare il consumo di suolo. Lo Stato deve investire in prevenzione, ma nella prossima legge di bilancio non c'è nulla sulla Carta geologica nazionale (CARG), né sulla cura del letto dei fiumi: la difesa del suolo non è in agenda. Non c'è il censimento degli edifici esistenti in riuso per il riutilizzo, i cui dati Istat sono aggiornati al 2012. Per l'azzeramento del consumo di suolo i dati Istat del 2023 sono preoccupanti. Poi ci si toglie la divisa della Protezione civile e tutto torna come prima, consumo di suolo e cementificazione compresi. Pertanto, per rispetto delle vittime passate presenti e per evitare vittime future, indossiamo tutti la divisa della prevenzione civile.

mi sembra doveroso intervenire. Mi viene a noia - come direbbero i toscani - essere qui oggi, in questo momento, per l'ennesima volta a commemorare delle vittime delle vittime che muoiono per l'assurdità del tempo: nel 2023 non si può morire per una pioggia (abbondante, ma pur sempre una pioggia). Allora è tutto vero, ha ragione il senatore Renzi quando dice che è stato un gravissimo errore e si sa chi ne porta la colpa - abolire la struttura di missione Italia sicura, che era stata istituita dal Governo Renzi. È giusto dare atto a chi ha fatto le cose, anche se di una maggioranza diversa, di averle fatte talvolta bene. è altrettanto vero che in queste ore c'è il solito gioco allo scaricabarile e che quella Regione ha gli stessi colori politici da cinquant'anni, da una vita, per cui nessuno si può scaricare la coscienza davanti a delle morti talmente ingiuste.

anche da chi scalda semplicemente la poltrona senza fare il lavoro che andrebbe fatto. Mi riferisco a quelle opere pubbliche di cui sappiamo, ma anche semplicemente alla pulizia dei tombini,

Signor Presidente, avrei desiderato intervenire su qualunque altro argomento, ma non sulla morte nella mia terra Toscana. Il cordoglio è anzitutto alle vittime di questa nuova tragedia nelle ore in cui il Governo e gli enti territoriali stanno lavorando per garantire un rapido ripristino della normalità, emerge in tutta la sua interezza la crescente tragedia che vede purtroppo il tessuto urbano, artigiano

da subito. Le risorse che dovranno necessariamente ristorare i danni non potranno essere disgiunte da quella prevenzione di cui troppo spesso si parla, ma che non riesce a concretizzarsi nella consapevolezza dei rischi e in una necessaria rivisitazione delle norme e anche degli enti, come il potenziamento dell'autorità di bacino. Si parlava prima dell'unità di missione, ma esistono anche strutture che sarebbero già in grado di operare subito in questo senso, se dotate di poteri e di risorse sufficienti. Voglio dire, infine, che ci ricordiamo delle vittime, ma è doveroso ricordare anche le persone grazie al cui lavoro non ci sono state più vittime e citerò il caso della RSA «Il Molino», nel Comune di Rosignano, dove, nel momento in cui purtroppo decedeva la signora Giovanna Innocenti, ottantatreenne ospitata all'interno della struttura, nel momento stesso in cui arrivava un'onda di piena,

agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile possiamo evitare di piangere un numero ancora più alto di vittime. La Lega farà tutto quanto possibile, insieme al Governo e agli enti locali, per superare anche questa drammatica situazione, che speriamo non capiti

da toscano prendo la parola in preda a un grande dolore per quello che è avvenuto nella mia Regione giovedì 2 novembre. L'alluvione di giovedì scorso ha colpito pesantemente il cuore della Toscana, ha colpito pesantemente la parte Ovest della provincia di Firenze, la provincia di Pistoia, tutta la provincia di Prato, ma ha colpito in maniera rilevante anche le province di Pisa, di Livorno e di Lucca e ha spezzato i cuori di centinaia di migliaia di toscani, perché tutti hanno sentito il bisogno, in quei momenti drammatici, di stringersi attorno alle famiglie più pesantemente investite

Permettetemi, ovviamente all'interno di un cordoglio che è uguale per tutte le vittime, di ricordarne in particolare due, perché queste due persone - due coniugi,

Questi coniugi si trovavano nel Comune di Lamporecchio a bordo di un'auto e cercavano di tornare alla loro casa, ma a un certo punto, in corrispondenza di un ponte,

li avevano colpiti, ovviamente privi di vita. Una tragedia nella tragedia, che dà la misura di quello che è accaduto in Toscana nei giorni scorsi. Insieme all'espressione di questo profondo cordoglio, vorrei esprimere la vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni e sono tantissimi. Ho passato i giorni scorsi a fare visita a famiglie che hanno la casa allagata, a imprenditori, artigiani e commercianti che hanno le loro officine, i loro laboratori e le loro aziende allagate o distrutte, accanto ai sindaci di tanti Comuni che sono stati colpiti, che vedono le infrastrutture pubbliche duramente messe alla prova. *(Brusio).* potrebbe interessare: senatori, colleghi, grazie; stiamo parlando di un'alluvione e di morti. Presidente)*. Ho passato queste ultime ore accanto alle persone che hanno subito danni, perché tutti si aspettano grande vicinanza dalle istituzioni. Anche i danni al patrimonio pubblico sono rilevantissimi, al di là delle frane e degli smottamenti. Ricordo soltanto il caso del Comune di Quarrata, dove due terzi della biblioteca comunale e 20.000 volumi sono andati completamente distrutti, perché i locali della biblioteca sono stati invasi dalle acque e sono ora totalmente irrecuperabili. quindi la vicinanza a tutte queste persone. Infine, rivolgo un sentimento di ringraziamento fortissimo per i soccorritori che si sono impegnati da subito nel portare conforto alle popolazioni, a chi era rimasto isolato e a chi rischiava. Un ringraziamento ai tantissimi volontari, soprattutto ragazzi, che - come ricordava il senatore Renzi - hanno fatto rivivere la memoria degli angeli del fango dell'alluvione del 1966. Sono stati migliaia i giovani che si sono messi a disposizione, che non hanno nemmeno atteso una chiamata, ma si sono presentati dove c'era bisogno di aiutare, senza che nessuno dicesse loro che dovevano esserci. Consentitemi di fare due auspici, chiedendo al Presidente due minuti per terminare il mio intervento. Il primo auspicio riguarda la richiesta che fanno tutte le persone con cui ho parlato in queste ore: c'è bisogno

ed enti pubblici totali e rapidi. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti. presenteremo emendamenti al disegno di legge di bilancio. Si tratta di centinaia di milioni di danni, non facciamone una questione di colore politico: questa battaglia deve vederci tutti uniti per la Toscana e per tutte le zone del nostro Paese che sono state colpite dai fatti di giovedì

Non dimentichiamoci che queste quattro storie hanno dietro realtà territoriali non considerate in questi anni. Noi ci siamo dimenticati del nostro territorio, l'abbiamo lasciato un po' troppo a se stesso. occhi le immagini dell'alluvione, quelle immagini tremende che poco ci toccano fino a che l'alluvione non viene a bussarci a casa nostra. Quando però ci bussa, ci rendiamo conto dei drammi e dei danni.

rischiavano di morire ai piani bassi. Mi riferisco ai presidi, quelle persone che controllavano il territorio e che oggi sono stati tolti: i cosiddetti presidi idraulici,

minimizzano il rischio idraulico. Penso che qui oggi sia fondamentale commemorare e ringraziare, ma soprattutto parlare di prevenzione e di educazione,

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 dicembre. Nella seduta di oggi saranno discussi i seguenti argomenti: interpellanza, con procedimento abbreviato, sulla situazione degli impianti siderurgici ex costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione; discussione del disegno di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la riunione del Parlamento in seduta comune alle ore 9,30, l'ordine del giorno della seduta di domani prevede, a partire dalle ore 11: seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2; dalla sede redigente, disegno di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge in materia di associazioni sindacali militari e delega revisione strumento militare; decreto-legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali; legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Giovedì 9 novembre sarà discusso il decreto-legge in materia di politiche di coesione e immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati. Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione del disegno di legge sulla disciplina della professione di guida turistica, collegato alla manovra di finanza pubblica. La settimana dal 20 al 24 novembre sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sui decreti-legge. L'Assemblea si riunirà, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22, se necessario, per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi e per il decreto-legge in materia di misure contro il caro-prezzi energia, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Nella settimana dal 28 al 30 novembre saranno discussi i seguenti decreti-legge: immigrazione e sicurezza, attualmente all'esame della Camera dei deputati; misure in materia economica e fiscale. Nella settimana dal 4 al 7 dicembre, con sedute senza orario di chiusura, saranno discussi il decreto-legge per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. In apertura della seduta di martedì 14 novembre saranno commemorate le figure dell'ex senatore Mario Tronti e del sociologo Francesco Alberoni. La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria è convocata, per procedere alla sua costituzione, martedì 14 novembre, alle ore 14. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, di autorizzare la 7a Commissione a discutere in sede deliberante, durante la sessione di bilancio, il disegno di legge sull'istituzione di un contributo stabile all'Istituto dell'enciclopedia italiana.

Signora Presidente, la questione è talmente delicata e complessa che merita l'attenzione dell'Assemblea e di tutti noi ed è per questa ragione che abbiamo presentato un'interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento. Signora rappresentante del Governo, oggi le rivolgerò alcune domande molto precise, nella speranza di avere le risposte che non abbiamo avuto dall'audizione

Le devo dire con molto rispetto, signora rappresentante del Governo, che ci saremmo aspettati oggi la presenza del ministro Fitto. Lo chiameremo in causa durante questo intervento. Credo che la sua presenza qui sarebbe stata un atto di correttezza nei confronti del Parlamento, perché così sembra che in qualche modo voglia fuggire dalla realtà *(Applausi)*, forse dalle proprie responsabilità, ma sicuramente da una vicenda sulla quale bisogna fare luce. luce. Prima di rivolgerle le domande, voglio fare una premessa. La vicenda dell'ex ILVA è il simbolo del fallimento del Governo nel campo delle politiche industriali. È la prova della mancanza di una strategia nazionale per il nostro Paese, che per continuare ad essere forte dal punto di vista economico ha bisogno di una nuova e vera politica industriale, dotata di una visione di cui nei vostri provvedimenti non c'è traccia. Tale mancanza sta arrecando un grave danno al nostro patrimonio industriale. Infatti, i provvedimenti finora adottati dal Governo per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto ne hanno in realtà aggravato la crisi, capovolgendo un percorso finalizzato alla ripresa dei livelli produttivi e occupazionali, alla decarbonizzazione, alla produzione e alla messa in sicurezza ambientale nel sito, ma non solo: gran parte delle misure finora adottate rispondono alle richieste di ArcelorMittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto e della tutela della salute e dell'interesse nazionale. Ancora, il decreto-legge che è stato approvato ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro a favore di ArcelorMittal, per garantire la liquidità dell'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore, senza che tali interventi abbiano prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva e occupazionale. E ancora, sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che avrebbe dovuto portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo, con un investimento di circa 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma. E ancora, a fronte dello stralcio dal PNNR del finanziamento di un miliardo di euro destinato proprio ad attivare la produzione del preridotto, il Governo non ha finora chiarito quali e quanti risorse saranno messe a disposizione tramite il Fondo di sviluppo e coesione. La situazione dell'ILVA è sotto gli occhi di tutti estremamente preoccupante e, per alcuni versi, drammatica. Proprio ieri le organizzazioni sindacali si sono rivolte al Presidente della Repubblica per segnalare la drammatica condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e la preoccupazione per la sicurezza sociale e la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una progressiva e successiva, ulteriore riduzione fino a 1,7 milioni. Allo stato attuale, in Acciaierie d'Italia (ADI) sono occupati 3.500 dipendenti, su un totale di 8.200, e continua il ricorso agli ammortizzatori sociali.

che salirebbero fino a 2,5 miliardi. Nel corso dell'audizione che si è svolta qualche settimana fa alla Camera - non è un mistero - il presidente di ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando dal punto di vista giudiziario, finanziario e societario e, come lei sa, in quell'occasione ha anticipato le sue dimissioni.

finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal Fondo di sviluppo e di coesione, ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Tale accordo confermerebbe il cambio netto della posizione del Governo in favore di ArcelorMittal, compresa l'intenzione di cedere al gruppo franco-indiano la quota pubblica.

di comprendere quali siano le condizioni e le prospettive di ADI e la strategia che si intende mettere in atto per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà fondamentale del Paese. Non solo: vorremmo sapere come riuscirete a garantire il ripristino dell'intervento previsto dal PNRR con le disponibilità del Fondo di sviluppo e di coesione, come intendete altresì rifinanziare tutte le misure le misure definanziate dal PNRR e se intendete mettere a carico delle spettanze della Regione Puglia una quota consistente degli interventi previsti per il sito. Si chiede ancora se intenda rimuovere il rinvio *sine die* degli interventi di ambientalizzazione del sito, tenuto conto del giudizio pendente presso la Corte di giustizia europea e, ancora, se sia intenzione del Governo favorire la dismissione di altri importanti impianti siderurgici in Italia, a partire da quello di Piombino, e quali iniziative si intendano adottare per fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti dell'ex ILVA di Genova, Cornigliano, Novi Ligure e Porto Marghera, dove si sono registrati anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio, nonostante le dichiarazioni fatte al riguardo. Signora rappresentante del Governo, ci aspettiamo che oggi il Governo dica parole chiare e faccia capire se sia di suo interesse - di tutto il Governo - di tutto il Governo - procedere alla cessione delle quote pubbliche di ArcelorMittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare la società pubblica al controllo del capitale di ADI. Questa vicenda, come ho detto all'inizio, è la dimostrazione del vostro fallimento nel campo delle politiche industriali. Noi non molleremo però la presa e continueremo a utilizzare tutti gli strumenti parlamentari per fare in modo che su questa vicenda si faccia chiarezza, si assumano gli impegni che noi avevamo chiesto di assumere quando si approvò il provvedimento sull'ex ILVA, proponendo anzitutto un tavolo di programma con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni con un collegamento reale al piano per il risanamento ambientale e la ripresa delle attività produttive. Voglio dire però, in conclusione, che questa vicenda è la dimostrazione

Insomma voi, pezzo dopo pezzo, state smantellando il patrimonio industriale del nostro Paese, ma noi non ve lo permetteremo e faremo di tutto perché questo non avvenga.

necessari. In premessa, tengo tuttavia a precisare che il ministro Fitto avrebbe voluto essere presente oggi in Aula, ma purtroppo un impegno istituzionale concomitante e improvviso glielo ha impedito. Mi preme anche riconoscere che il ministro Fitto non si è mai sottratto al confronto sui temi di sua diretta competenza. *(Brusio.

al fine precipuo di individuare le migliori soluzioni per garantire, attraverso un utilizzo efficiente e sinergico di risorse pubbliche, anche europee e private, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione e degli investimenti all'interno dell'impianto produttivo di Taranto, nonché il rilancio dell'attività produttiva, salvaguardando i livelli occupazionali. In questo senso, il *memorandum* è funzionale esclusivamente a individuare gli elementi e le condizioni ritenuti necessari dalle parti al fine di realizzare i sopramenzionati obiettivi senza che dallo stesso discendano obblighi giuridici specifici. giuridici specifici. Quanto al coinvolgimento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, anche dalle interlocuzioni con il socio privato di Acciaierie d'Italia SpA, occorre ricordare che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2012 di delega di funzioni, il predetto Ministro è titolare delle funzioni e delle attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. In relazione all'impianto siderurgico di Taranto, risulta pendente una procedura di infrazione oggetto del recente intervento normativo di cui al decreto-legge n. 69 del 2023. Inoltre, al predetto Ministro è stata delegata ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la coesione territoriale relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale, nonché il coordinamento dei programmi di intervento volti al superamento della crisi socio-economica ed ambientale nell'area di Taranto. In secondo luogo, come ha riferito il ministro Urso nel corso dell'audizione svoltasi sul tema il 26 ottobre dinanzi alla X Commissione della Camera dei deputati e alla 9a Commissione del Senato della Repubblica, il rilancio sostenibile dell'impianto ex ILVA di Taranto, ossia l'unica acciaieria italiana che produce acciaio primario comprendente tutto il ciclo produttivo dal minerale al prodotto finito, rappresenta una fondamentale area di intervento nell'ambito del piano siderurgico nazionale che il Governo intende impostare. Con specifico riguardo al piano industriale, è noto che durante il Governo Conte II è stato presentato un piano industriale con l'obiettivo di raggiungere una produzione di 8 milioni di tonnellate entro il 2025, di cui 5,7 da altoforno e il resto da processo elettrico. In particolare, in data 10 dicembre 2020 veniva sottoscritto l'accordo di investimento tra ArcelorMittal e Invitalia per una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto. L'accordo prevedeva, tra l'altro, un aumento di capitale di AM InvestCo Italy SpA, la società affittuaria dei rami d'azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per 400 milioni di euro con acquisizione da parte di Invitalia del 50 per cento dei diritti di voto della società, nonché a maggio del 2022 un aumento di capitale sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni da parte di ArcelorMittal, con conseguente acquisizione da parte di Invitalia del 60 per cento del capitale della società, subordinato ad una serie di condizioni sospensive connesse all'acquisto da parte della società affittuaria dell'impianto di Taranto che qui di seguito si riportano: modifica del piano ambientale esistente per tenere conto delle modifiche del nuovo piano industriale; revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto; assenza di misure restrittive nell'ambito dei procedimenti penali in cui ILVA risultava imputata nei confronti di AM InvestCo. Ebbene, nessuno dei temi sopra richiamati è stato affrontato dai precedenti Esecutivi, mentre il Governo Meloni, mediante due diversi provvedimenti legislativi, il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, è intervenuto per garantire la continuità aziendale e si è riservato di assegnare le risorse pubbliche previste solo solo all'esito di un percorso istituzionale che consenta di definire chiaramente gli impegni anche dei privati che gestiscono attualmente l'impianto produttivo. A tal fine, è stato richiesto alla società di presentare un nuovo piano industriale che preveda anche l'intervento di decarbonizzazione approvato dagli organi sociali e soprattutto asseverato da un *advisor* esterno che certifichi la sostenibilità economica ed ambientale. All'inizio di quest'anno è stata varata un'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'attuale affittuaria per complessivi 750 milioni, che ha visto Invitalia contribuire con 680 milioni e ArcelorMittal con 70 milioni. La volontà di salvaguardare la continuità aziendale dell'ex ILVA attraverso un disegno organico è stata confermata con il decreto-legge salva infrazioni, che ha neutralizzato ogni effetto ostativo all'acquisto dell'azienda, prevedendo che l'operazione possa legittimamente compiersi, pur in costanza di provvedimenti di sequestro e confisca eventualmente ancora esistenti sugli *asset*

al capitale della società in capo ad ArcelorMittal al 62 per cento, come già ricordato, a fronte del 38 per cento dello Stato tramite Invitalia. Quanto alla dotazione del Fondo di sviluppo e coesione e all'asserita decisione del Governo di porre a carico della Regione Puglia parte degli oneri finanziari relativi alla realizzazione degli interventi previsti per il sito, si rappresenta rappresenta preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, giusta le previsioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 144 del 2022, finanzia con un miliardo di euro la realizzazione nel sito di Taranto di un impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto (*direct reduce iron,* DRI). Tale intervento è strettamente connesso alla realizzazione del forno elettrico all'interno del medesimo impianto e alimentato mediante il preridotto. Senza la realizzazione del forno elettrico, dunque, l'impianto finanziato dal PNRR non avrebbe alcun senso, ne produrrebbe alcuna utilità. Quindi, la proposta del Governo di sostituire la fonte di finanziamento dell'intervento in questione è funzionale a garantire la realizzazione, evitando che la complessità della situazione connessa all'impianto di Taranto possa interferire con il il rigido cronoprogramma del PNRR, che - come è noto - prevede delle *milestone* e dei *target* stringenti, la cui osservanza costituisce la *condicio sine qua* *non* per la rendicontabilità della spesa e per l'erogazione delle somme da parte della Commissione europea. A tal fine, appare necessario ricordare che la decarbonizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto si ottiene non soltanto stanziando un miliardo per l'impianto DRI, ma anche realizzando forni elettrici e soprattutto assicurando all'acciaieria di Taranto un approvvigionamento di energia pulita nella quantità necessaria per assicurare il pieno funzionamento dell'impianto. Relativamente all'asserita decisione del Governo di porre a carico della Regione Puglia parte dell'onere finanziario relativo all'effettuazione degli interventi di decarbonizzazione dell'impianto, si evidenzia che non è stata assunta alcuna decisione di questo tipo. Vieppiù, alla luce della nuova disciplina relativa all'utilizzazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, delineata dall'articolo 1 del cosiddetto decreto Sud, si fonda sullo strumento pattizio degli accordi per la coesione. Quanto all'intervento di ambientalizzazione del sito si evidenzia che - come già rappresentato alla Commissione UE - nell'ambito della procedura di infrazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di giudizio l'AIA del 26 ottobre 2012 conteneva condizioni autorizzative immediatamente cogenti e significativamente più severe rispetto a quelle tipicamente poste alle altre installazioni, nonché ulteriori misure rispetto alla mera applicazione delle migliori tecniche poste a riferimento a livello comunitario, condizioni che hanno portato sin da subito a disporre il fermo degli impianti non adeguati ambientalmente. Come attestato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'attuazione di tali misure, tra cui limite legale alla produzione, adottate dapprima, conformemente all'AIA del 2012 e successivamente anche in conformità dei ministri del 2017, ha comportato già dal 2012 la riduzione delle emissioni provenienti dall'impianto siderurgico di Taranto e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell'aria, rilevato periodicamente dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. I dati, infatti, confermano che, con riferimento agli inquinanti monitorati dalla rete, la qualità dell'aria a Taranto rispetta i valori limite fissati dal decreto legislativo n. 155 del 2010, in conformità alla vigente direttiva europea 2008/50/CE. Con riguardo alle polveri fini, inquinante oggetto di prescrizioni AIA particolarmente rigorose, dalle rilevazioni emerge che nell'area circostante lo stabilimento i livelli di concentrazione sono inferiori non solo al valore limite imposto dalla normativa, ma anche rispetto ai livelli rilevati in altre aree della Regione Puglia. Con specifico riferimento all'attuazione degli interventi di adeguamento di cui al Piano ambientale del 2017, si rappresenta che dalle attività del cosiddetto osservatorio ILVA, nell'ambito delle quali sono stati acquisiti gli esiti delle attività di controllo effettuate dall'ISPRA, risulta che tutti gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

In merito ad alcuni interventi ambientali residuali, il raggiungimento degli obiettivi ambientali attesi è stato garantito dal gestore attraverso misure alternative agli interventi già previsti e in corso. Anche tali misure sono verificate da Ispra nell'ambito delle relative attività di controllo. Si evidenzia infine che attualmente gli impianti in esercizio del siderurgico di Taranto sono ambientalmente adeguati, ossia contengono gli interventi di adeguamento prescritti dal predetto decreto Relativamente all'istituzione di un tavolo permanente, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, finalizzato a fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti ex ILVA e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto, si evidenzia che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha già da tempo avviato interlocuzioni con le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali e di categoria per la definizione delle misure e delle azioni necessarie al superamento delle criticità, criticità socio-economiche e ambientali dell'ex ILVA di Taranto. [**Presidenza il 27 settembre a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'ex ILVA di Taranto, alla quale hanno partecipato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto. In questa circostanza il Governo ha ribadito la consapevolezza dell'urgenza degli interventi e l'impegno a dare soluzioni di prospettiva, concentrando la propria azione in modo prioritario sul completamento del percorso di decarbonizzazione, sulla positiva definizione delle procedure di infrazione in atto, sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell'impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti. Successivamente, il 20 ottobre, si è svolto un nuovo incontro con i sindacati FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM per fare il punto sulle principali criticità che interessano gli impianti di produzione. In tale occasione è stata definita una *road map* nel confronto in corso con l'azienda, con due confini invalicabili

ossia l'impianto ex ILVA di Genova Cornigliano; Terni, per il quale l'obiettivo è un consolidamento dell'ottimo lavoro svolto nel corso della precedente legislatura dal ministro Giorgetti per il rafforzamento della produzione di acciai speciali (proprio per illustrare le prospettive di crescita dell'impianto, il ministro Urso, nel corso dell'audizione del 26 ottobre, ha comunicato di aver convocato una riunione con le organizzazioni sindacali per il prossimo 14 novembre); impianto che possiede enormi potenzialità, in particolare sulle rotaie. Si tratta di una caratteristica particolarmente interessante nell'ottica dello sviluppo del mercato interno, nonché del mercato europeo e di quello del bacino del Mediterraneo. Proprio per tali motivi il ministro Urso, nel corso della citata audizione, ha comunicato di aver fissato, per il prossimo 8 novembre, un incontro con i sindacati dei lavoratori dello stabilimento, per illustrare le prospettive di sviluppo del polo di Piombino.

far convivere stabilimenti complessi nei decenni che abbiamo alle spalle. Sono città che hanno dato un contributo straordinario al nostro Paese. Signor Presidente, la vicenda di Acciaierie d'Italia... Capisco che a molti possa non interessare il destino di migliaia di lavoratori. PRESIDENTE. No, interessa. Prosegua, abbiamo richiamato l'Assemblea proprio per questo. E soprattutto mi pare di capire che, di fronte alla fuga del ministro Fitto dalle sue responsabilità, la maggioranza non senta nemmeno il sentimento delle scuse verso i lavoratori. Non è la prima volta, purtroppo è già accaduto. Signor Presidente, ci saremo aspettati dalla Sottosegretaria una risposta chiara alle domande che il senatore Martella le ha posto; ma lei ci ha risposto ricordandoci le deleghe del ministro Fitto. Francamente non ne sentivamo il bisogno. Non mi pare che abbia firmato un *memorandum*, che ancora oggi è sconosciuto al Parlamento, per procedura di infrazione, perché, se così fosse, lo avrebbe potuto rendere visibile a tutti. Non ci pare che abbia firmato un *memorandum* per le sue deleghe sulle politiche di coesione.

e lo ha prelevato esattamente come si faceva nel periodo 2008-2011 con il FAS, il Fondo per le aree sottoutilizzate, che veniva utilizzato come Bancomat per svuotare il Mezzogiorno. Questa volta - lo dico ai colleghi del Mezzogiorno della maggioranza - lo sport del Governo Meloni è far diminuire le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione. Allora, signor Presidente, vogliamo che resti a verbale una cosa molto chiara: noi non ci fermeremo qui. I lavoratori hanno scritto al Presidente della Repubblica. Noi li abbiamo incontrati nelle audizioni che abbiamo dovuto fare perché la manovra non arrivava. E quello che preoccupa tutti è che questa azienda, che nel 2013 produceva più di sei milioni di tonnellate, puntualmente, ogni volta che c'è stata una mediazione negli ultimi mesi sul piano industriale,

il senatore Martella ha rivolto alla Sottosegretaria quesiti che non hanno ricevuto una risposta. Noi oggi vogliamo sapere se la strada che abbiamo di fronte è quella dell'interlocuzione con il Governo o della denuncia delle omissioni del Governo agli altri organi di controllo. Noi pensiamo che sia molto grave aver firmato quel *memorandum*. Ricordiamo le contestazioni fatte dall'amministratore delegato di Invitalia ad Acciaierie d'Italia, cioè la mancata comunicazione al socio pubblico in merito allo stato della società siderurgica sul possibile esercizio dei propri diritti. È necessario dare risposte chiare rispetto ai flussi di cassa a dodici mesi per far fronte all'impegno assunto di portare la produzione di acciaio a quattro milioni di tonnellate e non sappiamo meno rispetto ai nuovi patti che sono stati sottoscritti. Infine chiediamo con forza, signor Presidente, al Governo se intende chiarire il futuro di Acciaierie d'Italia. Noi chiediamo che torni pubblica. Noi chiediamo che si facciano le verifiche su tutti gli scambi infragruppo da Acciaierie d'Italia d'Italia al gruppo Mittal, perché abbiamo la sensazione che i numeri non tornino. E se è così, signor Presidente, il Partito Democratico - e immaginiamo buona parte delle altre opposizioni - non si fermerà di fronte a questa fuga del ministro Fitto. Insisteremo Insisteremo fino a richiedere eventualmente una nuova amministrazione straordinaria. Non ci convince il percorso indicato da Fitto: o

azioni di sindacato ispettivo, attraverso indagini che inevitabilmente dovranno essere fatte rispetto all'utilizzo del Fondo di sviluppo e di coesione, attraverso gli interventi alla Corte dei conti. Vogliamo capire perché a un certo punto il Governo Meloni ha smesso di sostenere questa azienda con le aziende dello Stato e con la responsabilità diretta dello Stato e si è messa direttamente è messa direttamente - non ascoltando più i lavoratori, non ascoltando più il territorio, non ascoltando più le amministrazioni locali, non ascoltando più Regione Puglia - nelle mani del socio privato che ancora oggi e lo sottolineo nuovamente - non dà informazioni chiare sullo stato dell'azienda, che a noi pare essere in grave difficoltà nonostante il quadro commerciale, nonostante il quadro economico generale.

casi il ministro Giorgetti e il ministro Urso, rispetto alla responsabilità del ministro Fitto, si sono lavati le mani. La risposta di oggi è la conferma della fuga del Governo Meloni dalle responsabilità sulla vicenda delle ex Acciaierie ILVA, oggi Acciaierie d'Italia, e sul futuro degli stabilimenti di Taranto, Cornigliano, Novi Ligure e tutti gli altri stabilimenti citati dal senatore Martella nell'interpellanza urgente.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione. Il 25 ottobre 2023 il Consiglio di Presidenza ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea del Senato un intervento adesivo al ricorso presentato il 28 febbraio 2023 dalla Camera dei deputati dinanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Il conflitto in questione si riferisce alle sentenze,

della Camera dei deputati in ordine al contenzioso riguardante le procedure per l'affidamento degli appalti della Camera dei deputati. Con ordinanza n. 179 del 6 luglio 2023, depositata in cancelleria il 28 luglio 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso della Camera dei deputati e ha disposto la notifica dell'ordinanza stessa al Senato della Repubblica «stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni

nel considerare sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall'amministrazione della Camera, abbiano leso la sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli articoli 64, primo comma, e 55 e seguenti della Costituzione, che attribuiscono alle Camere «specifiche funzioni e una posizione di particolare indipendenza». Se non vi sono richieste di intervento, simultaneo della proposta del Consiglio di Presidenza di intervenire nel giudizio a fianco dell'altro ramo del Parlamento.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2***

Signor Presidente, prima di iniziare a svolgere la relazione, voglio ringraziare i membri della 10ª Commissione e il presidente Zaffini per come sono stati condotti i lavori, che sono stati impegnativi e lunghi, con una lunga discussione su un numero molto cospicuo di emendamenti e di ordini del giorno. È stato un lavoro positivo e proficuo. Il disegno di legge il titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è diretto a istituire e disciplinare una Commissione parlamentare d'inchiesta di carattere bicamerale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalle diffusione del virus SARS-CoV-2. Il provvedimento costa di sette articoli ed è stato oggetto di un ampio ed approfondito esame in Commissione. Il disegno di legge, inizialmente assegnato alla 10ª Commissione in sede redigente, a seguito della richiesta di rimessione all'Assemblea, formulato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, ha proseguito il proprio *iter* in sedere referente. Complessivamente, sono state svolte nove sedute. L'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera, prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità. Con un emendamento approvato in Commissione è stato previsto che, oltre alla prontezza ed all'efficacia, si debba valutare anche la resilienza di tali misure. Entro la fine della corrente legislatura la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Ai sensi dell'articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che facciano parte di quest'ultima quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche dei compiti assegnati alla Commissione e sono chiamati, entro dieci giorni dalla nomina, a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta. In base al comma 2, la convocazione per la costruzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato. Nel corso dell'esame in Commissione è stata approvato un emendamento che ha ampliato da dieci a quindici giorni il termine previsto per la predetta convocazione. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da due segretari ed è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due Vice Presidenti, come per quella dei due segretari, ciascun Commissario ha a disposizione un solo voto e risultano eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti. L'articolo 3, che definisce in modo puntuale i compiti della Commissione di inchiesta, è stato modificato da diversi emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione. In particolare, è stata eliminata la previsione contenuta alla lettera che contemplava, tra i compiti elencati dalla norma, la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. A seguito delle predette modifiche in sede emendativa, i compiti attribuiti alla Commissione d'inchiesta riguardano: la valutazione dell'efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e dell'impatto del SARS-CoV-2, l'esame dei documenti, dei verbali, degli scenari di previsione e dei piani da esso eventualmente elaborati o sottoposti alla sua attenzione: lettere *a)* e *b)*; l'accertamento delle vicende relative al piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia da influenza (cosiddetto piano pandemico), del mancato aggiornamento del piano redatto nel 2006, della mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza il 3 gennaio 2020, e delle ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo e al suo mancato aggiornamento; nonché l'accertamento dell'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al virus SARS-CoV-2 (lettere *c*, *d*, la verifica dei compiti e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della *task force,* istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020, incaricata di coordinare le iniziative in tema di Covid-19 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (lettera *g*); la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il Regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi (lettera l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, gli organismi dell'Unione europea - quest'ultimo è un riferimento introdotto da un emendamento approvato in Commissione - e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettera *i*); l'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito Internet dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera la valutazione della tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica (lettera la valutazione della tempestività e dell'adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e distribuiti alle Regioni nel corso dell'emergenza (lettere *n* ed la verifica sull'esistenza di eventuali carenze o ritardi nell'approvvigionamento dei beni appena citati e l'individuazione delle relative cause e responsabilità (lettera *p*); l'indagine su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per la protezione dai contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e nel corso della pandemia (lettera *q*); l'indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità o illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento e alla cura del Covid-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del commissario straordinario, tra i quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da Covid-19 e degli *hub* vaccinali tra cui centri temporanei di vaccinazioni denominati "Primule", la realizzazione dell'applicazione "Immuni", la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni (lettera la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia verificando il fondamento scientifico delle stesse anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta e i risultati ottenuti da altri Stati europei (lettera Tale previsione è stata oggetto di modifica in sede emendativa, eliminando il riferimento a eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali. la verifica del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle misure di contenimento adottate (lettera *u*); la valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate dal Governo per la prevenzione e gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali la verifica dell'efficacia, adeguatezza e congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo la verifica dell'eventuale conflitto di interessi tra i componenti degli organi tecnici governativi, delle associazioni di categoria e delle case farmaceutiche (lettera *bb*); la verifica dell'efficienza e della corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure dei soggetti più fragili (lettera *cc*); l'indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia, nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto, come precisato a seguito di un emendamento approvato in Commissione, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili (lettera la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) precedenti all'autorizzazione dell'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera *ee*); la stima e la valutazione dell'incidenza, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possano aver avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per Covid-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi postvacciniche denunciate L'articolo 4 disciplina poteri e limiti della Commissione. In primo luogo, essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; non può, peraltro, adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione, nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per l'audizione a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale. Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non possono essere opposti il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della legge L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione d'inchiesta; nel testo trasmesso dalla Camera si prevede la possibilità per quest'ultima, nelle materie attinenti alle finalità del provvedimento, di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti relativi a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, nonché di atti e documenti custoditi da organi e uffici delle Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento che ha limitato la possibilità di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ai soli atti non coperti da segreto di indagine. La disposizione prevede inoltre il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Fermo restando tale vincolo, spetta alla Commissione stabilire quali atti o documenti sono coperti dal segreto e comunque non devono essere divulgati anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto in esame siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari d'inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. L'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti d'inchiesta segretati. La violazione di tali obblighi e la diffusione di tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. L'articolo 7 demanda la disciplina delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno da approvare prima dell'avvio dell'attività di inchiesta. La Commissione può organizzare i propri lavori anche mediante uno o più comitati; si riunisce normalmente in seduta pubblica, ma ha facoltà di riunirsi in seduta segreta qualora lo si ritenga opportuno; può avvalersi dell'opera di agenti ufficiali della polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessario di soggetti interni o esterni alle amministrazioni dello Stato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dei Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Per il suo funzionamento è stabilito un limite di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2023

allo svolgimento dell'inchiesta. La Commissione, infine, è chiamata a curare l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Vorrei anche ricordare alle colleghe e ai colleghi in quest'Aula che sarebbe davvero utile da parte di tutti quanti noi fare una sorta di passo indietro con la memoria quando parliamo del Covid, della pandemia, di quello che è successo nei primi mesi del 2020. Vorrei anche che ricordassimo il senso di smarrimento, la paura che in qualche modo era e fu in quei giorni un sentimento di tantissimi, io credo del tutto naturale. Vorrei anche che provassimo a immedesimarci in tutte quelle persone che poi quell'emergenza hanno dovuto effettivamente affrontare e soprattutto chi doveva prendere delle decisioni: il presidente del Consiglio Conte, il ministro della salute Speranza innanzitutto,

di chi prese quelle decisioni in una condizione molto difficile e dolorosa per il Paese, avendo peraltro a disposizione - ricordiamolo tutti - pochissime informazioni perché, soprattutto all'inizio, all'inizio, nella primissima fase del Covid, anche semplicemente accedere alle informazioni non era una cosa facile. Ricorderete anche, Presidente - se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io - che le attuali forze di Governo in quel momento erano all'opposizione e si contraddistinsero per una serie di vere e proprie speculazioni politiche. L'attuale Presidente del Consiglio, in quei mesi, in quei momenti, era contraria alla proclamazione dello stato d'emergenza. Vorrei anche ricordare gli indimenticabili video del ministro Salvini, che un giorno chiedeva l'apertura di tutto e il giorno dopo chiedeva la chiusura di tutto. Davvero non voglio immaginare cosa sarebbe successo se al posto

a votare l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su quel periodo e sulla gestione della pandemia e - come dicevo

se la legge istitutiva l'avesse delegata a svolgere un'indagine seria sul sistema del Servizio sanitario nazionale e regionale per capire, per esempio, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato; come modificare eventualmente il Sistema sanitario per renderlo più efficiente, anche nel caso malaugurato in cui dovessimo nuovamente trovarci dinanzi a un'emergenza come fu quella, e per valutare, per esempio, se la regionalizzazione della sanità, con la quale ormai ci confrontiamo da molti anni, sia stata utile oppure - come fu durante i mesi della pandemia - sia stata drammaticamente dannosa. Penso che la maggioranza di Governo la risposta la stia dando già nel corso di questi mesi. mesi. Quando pensa di voler costruire un provvedimento come quello sull'autonomia differenziata, in realtà ci sta dicendo che quella regionalizzazione è giusta ed è corretta. Io penso evidentemente il contrario penso che oggi sarebbe corretto fare una valutazione di merito molto più attenta di quella meramente propagandistica che viene portata avanti. Questo disegno di legge istitutivo in realtà assegna alla Commissione d'inchiesta un compito molto diverso da quello che ho appena ricordato, ho appena ricordato, ossia costituire un vero e proprio processo politico, un inaccettabile processo politico *(Applausi),* contro chi in quegli anni era al Governo e, per l'appunto, ha provato a contrastare la pandemia. Avete delimitato il perimetro dell'indagine e avete tenuto fuori deliberatamente - sono stati presentati molti emendamenti in tal senso - i Governi delle Regioni. Non è particolarmente difficile immaginarne il motivo, visto che le Regioni che hanno avuto le gestioni più critiche erano guidate dalle forze politiche dell'attuale maggioranza, una per tutte la Lombardia. Voi davvero pensate che si possa fare una seria indagine sull'emergenza pandemica escludendo dall'analisi la situazione dei Servizi sanitari regionali e le decisioni che furono prese a livello regionale? Davvero il tasso di strumentalità deve arrivare a questo? Io credo che sia davvero sufficiente questo per dimostrare che non vi interessa una Commissione che indaghi seriamente e che l'obiettivo politico, anche della discussione che stiamo facendo stasera, è un altro. Il punto però, Presidente, oltre a queste

con la natura stessa dell'istituto della Commissione, che rappresenta un potere strumentale del Parlamento, che ha il fine di condurre a riforme e a nuove proposte legislative e che eventualmente può avere la funzione di indirizzo verso il Governo. Non lo dico io, ma la Corte costituzionale, che lo ribadisce che compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è quello di giudicare,

con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso»; di tale delicato e necessario Nel caso odierno in discussione, l'obiettivo è un vero e proprio nuovo processo. Non contenti peraltro delle archiviazioni che già ci sono state da parte della magistratura, la pretesa è nuovamente quella di processare gli avversari politici, senza alcun rispetto delle prerogative della stessa magistratura e soprattutto senza alcun rispetto del diritto alla difesa delle persone coinvolte. Ricorderete che recentemente lo stesso presidente Mattarella, durante la cerimonia del ventaglio dello scorso luglio, ha sottolineato l'assoluta necessità del rispetto della separazione dei poteri. Ha detto testualmente che ciascuna istituzione deve fare la sua parte, rispettando l'ambito di attribuzioni affidate agli altri poteri, sottolineando come le iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre l'attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate. Non esiste, cioè, un contropotere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio ancora, in conflitto con l'azione della magistratura. Eppure, avete deciso di andare avanti,

che assegna - come sappiamo bene - un ruolo determinante e chiare competenze alle Regioni in materia sanitaria. Questo disegno di legge, dal nostro punto di vista, contrasta proprio con perché non tiene in alcun conto il disposto di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, che prevede in capo alle Regioni il potere di introdurre ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste, per far fronte a sopravvenute situazioni specifiche di aggravamento del rischio sanitario. Insomma, a me pare evidente che, dinanzi a questa indiscutibile competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione e nell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, qui si stia procedendo in tutt'altro modo, per una evidente ragione politica, strumentale, cinica e propagandista. *(Applausi)*. Siccome poi per

una crociata contro il vaccino, quello che si è nutrito del peggior complottismo e del peggior negazionismo, quello che abbiamo visto all'opera nel corso degli anni scorsi. *(Applausi)*. Ecco, forse lo fate perché dovete parlare a loro, perché dovete parlare a quelle persone. Credo davvero che la discussione di stasera offenda tutti quanti noi e penso soprattutto che sia profondamente contraria alla nostra Costituzione. È per questa ragione che vi chiediamo di non procedere all'esame del provvedimento.

il testo che dovremo analizzare e che io mi auguro invece venga respinto da quest'Assemblea, alla fine di questa discussione sulla pregiudiziale, in realtà pone un tema che appartiene a tutti Ci appartiene perché presenta un tema fondamentale per la tutela della salute, la tutela della salute, che non riguarda solamente la legge che viene istituita dallo Stato, ma istituita dallo Stato, ma riguarda specificatamente una materia che è definita *shared competence* tra lo Stato e le Regioni. Questo è definito dall'articolo 117 della Costituzione. A me pare molto superficiale il fatto che alcuni onorevoli colleghi senatori non tengano in debito conto la Costituzione italiana. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del virus come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, l'11 marzo 2020, è stata riconosciuta dall'OMS una situazione pandemica. Il Governo, di fronte a questa situazione pandemica, ha dichiarato lo stato d'emergenza.

sempre citata questa intesa con la Regione? Perché qualsiasi materia in questo campo deve essere discussa anche con la Regione; quindi anche la Regione aveva una voce in capitolo. Tutti ci ricordiamo all'inizio quel mosaico di decisioni che sono state prese dalle Regioni. Se ve lo ricordate - io lo ricordo bene alcune Regioni remavano anche contro le decisioni che venivano prese dal Governo. *(Applausi)*. Una di queste Regioni - lo ha ricordato già il mio collega De Cristofaro - era la Lombardia, dove c'è stata la maggior parte dei morti

nella Regione che ha avuto il maggior numero di morti. Che significa questo realmente? Significa dare la possibilità ad una Commissione parlamentare di manipolare la verità.

escludendo tutti gli enti territoriali, e in particolare le Regioni, da questa indagine. a noi ingiustificabile non è solamente questo atteggiamento di ostruzionismo nei confronti di un'indagine. Appare veramente ingiustificata la superficialità con cui si vuole affrontare questo argomento, che riguarda, lo ripeto, un interesse pubblico. Questo riguarda anche l'articolo 82 della Costituzione sulla istituzione della Commissione parlamentare,

È questo il motivo e siete voi che state nascondendo la verità ai cittadini italiani. Ci sono giovani cittadini italiani che ci stanno guardando.

e questa Commissione parlamentare d'inchiesta, a costo di ripetermi, non rispetta la Costituzione italiana, perché ne vìola gli articoli 117 e 82. Vorrei anche 82. Vorrei anche entrare nel merito di una sentenza costituzionale che è stata citata anche da un mio collega, proprio per ribadire quanto sto dicendo. Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975 ha affermato che compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è quello di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio della funzione delle Camere. E qual è questo esercizio? Raccogliere materiale di pubblico interesse. Ritorniamo al pubblico interesse. È un cortocircuito quello che si sta realizzando con questa Commissione parlamentare d'inchiesta. Nella percezione pubblica vorrei ricordarvi la locuzione "gestione dell'emergenza epidemiologica". Cosa ci dice tale locuzione? Qualcuno me lo sa dire? Significa definire un perimetro temporale. Non si può fare epidemiologia, e questo i medici che sono in Aula lo dovrebbero sapere, senza definire un periodo temporale.

In poche parole, questa Commissione nasce monca, incapace di appurare la verità dei fatti e l'avete costruita in questo modo per nascondere la verità *(Applausi)* e cioè che le Regioni che avete amministrato non sono state in grado di gestire la pandemia. È per questo motivo, signor Presidente, che noi vogliamo che si deliberi di non procedere all'esame del testo unificato del disegno di legge n. 790, anche perché questo svilisce e travisa un istituto prezioso come la Commissione d'inchiesta.

Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici,

le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità. Nello svolgimento di tale compito, la Commissione di inchiesta dovrebbe analizzare e valutare le misure adottate dal Governo nel corso dell'emergenza epidemiologica. Dovrebbe inoltre valutare le condotte tenute da organismi internazionali e sovranazionali, quali l'OMS, nonché quali l'OMS, nonché la Commissione europea e l'Agenzia europea per i medicinali, nonché ancora gli atti del procedimento di revisione continua dei vaccini anti-SARS.

dalle Regioni nell'organizzazione dei servizi sanitari e, più in generale, nell'azione di contenimento della pandemia. Dunque l'oggetto e il perimetro di questa Commissione d'inchiesta prevedono una valutazione e un'analisi degli atti compiuti dal Governo e una valutazione e un'analisi degli atti compiuti da soggetti internazionali, ma escludono espressamente qualsiasi valutazione nei confronti degli atti e dei comportamenti tenuti dalle Regioni e dalle articolazioni regionali che strutturano il nostro Servizio sanitario nazionale. Quali siano, onorevoli colleghi, le ragioni di una simile esclusione è assai difficile da capire.

al di fuori del perimetro costituzionale di cui all'articolo 82 della Costituzione. Come ha infatti affermato la Corte costituzionale già dalla fondamentale sentenza n. 231 del 1975, il compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta dovrebbe essere quello di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso. lasciare l'attività delle Regioni del tutto al di fuori del perimetro dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta impedisce di verificare innanzitutto l'impatto negativo della frammentazione dei sistemi sanitari regionali di fronte a emergenze massive come la pandemia; impedisce inoltre di verificare se e in quale misura abbiano inciso sulla concreta gestione dell'emergenza pandemica scelte di politica sanitaria operate in precedenza e rivolte, ad esempio, a indebolire la sanità territoriale e le cure di prossimità, favorendo l'ospedalizzazione; e impedisce altresì di avere un quadro preciso delle effettive necessità dei sistemi sanitari regionali anche sul piano finanziario e di articolare con il necessario equilibrio il bilanciamento tra decentramento delle politiche sanitarie e garanzie di istanze unitarie, particolarmente evidenti e rilevanti proprio nel caso delle emergenze di carattere nazionale. L'obiettivo dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta dovrebbe essere quello di indagare, in spirito di leale collaborazione istituzionale e di concordia politica, sulla funzionalità e sulla resilienza complessiva del sistema, di fronte a una situazione straordinaria quale quella determinatasi in conseguenza della pandemia, individuando punti di forza e punti di debolezza, al fine di consentire al Parlamento e al Governo di articolare politiche volte a rafforzare la sanità e a garantire piena e uguale tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, sia sul piano del potenziamento delle strutture di prossimità, sia al fine di aumentare e meglio impiegare le risorse del sistema nazionale e di quelli regionali. L'accertamento delle modalità di azione delle Regioni infatti, in questa prospettiva, è fondamentale per verificare proprio l'efficacia e l'effettiva resilienza delle misure complessivamente adottate per il contrasto dell'emergenza pandemica, anche e soprattutto con riferimento a specifiche situazioni critiche verificatesi in alcuni sistemi sanitari regionali, come ad esempio quello lombardo, e con lo specifico fine di individuare la necessità di interventi volti a superare carenze strutturali e sistemiche dei sistemi sanitari regionali e di quello nazionale. Tale esclusione, onorevoli colleghi, è davvero priva di qualsiasi giustificazione, tanto più se noi consideriamo come nel corso dell'emergenza siano stati assunti da parte delle Regioni, in collaborazione con il Governo, una pluralità di atti amministrativi, a conferma del fatto che il ruolo delle Regioni, delle amministrazioni regionali e delle articolazioni amministrative del Servizio sanitario nazionale a livello regionale è stato assai significativo e, in molti casi, determinante. Se si vuole trarre un qualche insegnamento da ciò che è accaduto, dalla tragedia che si è consumata e dalle tante morti che purtroppo si sono verificate durante la pandemia, allora bisogna evitare qualsiasi strumentalizzazione; bisogna avere un atteggiamento costruttivo e intellettualmente onesto che cerca di approfondire tutti gli aspetti di quella complicata vicenda.

quale sia stato il ruolo delle Regioni e quali siano state le loro carenze, non sempre per responsabilità delle amministrazioni regionali, ma per l'assetto complessivo, che andrebbe

e sugli atti cosiddetti emergenziali del Governo. A che fine? È evidente che i risultati saranno parziali. È evidente che non potranno emergere le carenze o invece i punti di forza della reazione alla pandemia. È quindi evidente che stiamo - anzi, state - per approvare un atto inutile, per non dire dannoso. Infatti, alla fine, riaprire su terreni una polemica tra detrattori dell'obbligo vaccinale e fautori della necessità di adottare con responsabilità tutte le misure che la scienza suggerisce di adottare non porterà molto lontano e io temo che non farà un gran servizio al nostro Paese, che avrebbe invece bisogno - lo ripeto - di guardare a quella tragica vicenda con occhi più equilibrati e con l'intenzione di trarne un insegnamento, affinché le tante, troppe carenze del Servizio sanitario nazionale non abbiano in futuro a ripercuotersi sui cittadini più fragili.

a pochi giorni dall'approvazione di questo disegno di legge alla Camera, il Presidente della Repubblica ha speso parole molto chiare: «Iniziative di inchiesta con cui si intende sovrapporre l'attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate. Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l'azione della magistratura. come non sono le Camere a poter verificare, valutare e giudicare se norme di legge, che il Parlamento stesso ha approvato, siano o meno conformi alla Costituzione, perché questo compito è riservato dall'articolo 134 in maniera esclusiva alla Corte costituzionale». Sulla scorta di queste parole, il Senato ha apportato alcune modifiche al testo approvato dalla Camera, ma a nostro avviso queste non bastano per soddisfare le obiezioni sollevate dal Presidente della Repubblica. L'articolo 3 della legge continua ad assegnare a questa Commissione un campo enorme di funzioni e compiti, con un allargamento a campi che non sono di sua competenza, che rischiano di ingenerare un vero e proprio cortocircuito tra poteri dello Stato. La Commissione infatti assume, tra i compiti in elenco all'articolo 3, quello di valutare, ossia di esprimere un giudizio di merito, ad atti e fatti. Tutto questo è in palese contrasto con quanto sancito dalla sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, la quale afferma che compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è giudicare, ma solo raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere o per invitare il Governo ad adottare i provvedimenti del caso. Le funzioni della Commissione sono un concentrato di tesi precostituite, tesi che per l'intera stagione del Covid sono state l'armamentario propagandistico dei partiti che all'epoca sedevano all'opposizione. Lo scopo politico emerge anche dalla volontà di limitare l'ambito di indagine agli ultimi due Governi, escludendo cioè tutti quegli enti locali, a partire dalle Regioni amministrate dal centrodestra, che hanno avuto un ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza pandemica. Una Commissione d'inchiesta sul Covid avrebbe dovuto riportare all'articolo 3 un semplice rigo: indagare le criticità emerse per aiutare il decisore pubblico nella riflessione sulle politiche e gli strumenti da sviluppare per la gestione di eventuali nuove pandemie. Questo a chi ha promosso la Commissione sembra non importare. La sofferenza e il dolore che hanno patito l'Italia e il mondo intero vengono usati come clava per colpire gli avversari politici: nulla di più sbagliato. Il Gruppo per le Autonomie voterà quindi a favore delle pregiudiziali di costituzionalità.

Ciò chiamerebbe ad una riflessione sul fatto che voi state discutendo e volete imporre l'autonomia differenziata, quando il vero fallimento è la regionalizzazione della sanità, questo è il dato fondamentale. Al riguardo anche il centrosinistra deve fare una riflessione, perché questa regionalizzazione non ha portato un miglioramento della sanità, ma un peggioramento rispetto alla legge n. 833 del 1978. Anziché avere un sistema unico e universale, ha portato a una frammentazione. Vogliamo discutere francamente di questo problema?

su questo, perché abbiamo pensato che, anziché avere un sistema sociosanitario assistenziale, avevamo un'azienda: la sanità è diventata un'azienda e, se è un'azienda, deve fare profitti, non *(Applausi)*. Questo è ciò che è avvenuto. Allora discutiamo, facciamo l'inchiesta, ma proviamo tutti a ragionare con grande umiltà di questi problemi e cerchiamo di dare qualche risposta in merito. Se vogliamo discutere delle responsabilità di ogni Regione, riguarda la Val Seriana, dove non c'è paese in cui una famiglia non abbia avuto un morto, la responsabilità sarà di Conte e di Speranza o di tutti quelli che erano lì, a partire dagli imprenditori che hanno detto che non si dovevano chiudere le aziende? La diciamo questa cosa, la facciamo questa discussione o ne

il signor Fontana e i leghisti non c'entravano niente, visto che hanno la maggioranza da una vita in quel territorio? Oppure Gallera, che si è dovuto dimettere per incapacità e che avete poi rieletto? *(Applausi)*. Ma di che cavolo vogliamo parlare?

perché la storia su questo vi sconfiggerà, punto. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo essere molto onesti intellettualmente, espressione che ha utilizzato un collega che stimo, il senatore Giorgis, e affrontare il tema che va affrontato, che non è un comiziaccio vecchia maniera sulle responsabilità dell'impresa, che va bene per un discorso sindacale, non per una pregiudiziale di costituzionalità, ed entrare nel merito: noi domani spiegheremo perché è giusto votare sì all'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, come abbiamo votato sì all'istituzione delle Commissioni di inchiesta nelle Regioni, a cominciare dalla Lombardia. Oggi siamo a ragionare di tre questioni pregiudiziali, la cui esposizione da parte del collega De Cristofaro, del collega Mazzella e del collega Giorgis ho ascoltato con grande interesse, quale sia il motivo costituzionale per cui questa Commissione non s'ha da fare. C'è poi un elemento che affronteremo domani e cioè perché si debba istituire o meno la Commissione, ma qui siamo su un principio di diritto, l'articolo 82 della Costituzione, che consente alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, ponendo come unico limite non travalicare senatore De Cristofaro per il tramite del Presidente del Senato: vi rendete conto che avete chiesto di bloccare una Commissione d'inchiesta in nome di un principio costituzionale dopo che ne abbiamo fatte 97 in questo Parlamento?

Mi si dice - e lo dice bene il senatore De Cristofaro, altro collega che stimo, pur non condividendone le opinioni - di pensare cosa sarebbe accaduto se fosse stato Primo Ministro Salvini. è un tema politicamente rilevante: io, pur di mandare a casa Salvini - e il collega De Cristofaro lo sa - ho anche fatto l'accordo con i Cinque Stelle, contestato dal centrodestra; si immagini se non sono sensibile all'argomento. Questo però con la Costituzione che c'entra? Il collega De Cristofaro Il collega De Cristofaro dice che diamo spazio ai no vax. A me lo dice il collega De Cristofaro? Chiedetelo alla senatrice Lorenzin, che è stata Ministro del mio Governo, che ha fatto un decreto sui vaccini, quando non c'era la pandemia all'orizzonte, contestatissimo. Chiedetelo a noi, che abbiamo invitato Roberto Burioni a una Leopolda; chiedetelo a me, che ho chiesto a Burioni di candidarsi nel 2018. A me lei viene a parlare di vaccini? Che ci azzecca con la Costituzione? Voi avete posto una questione politica, che è legittima, ma non c'entra niente con la Costituzione. Il senatore Mazzella dice che vorrebbero sapere cos'ha fatto il presidente De Luca, che è un tema affascinante, perché siamo in tanti a domandarci, in generale, che cosa farà il presidente De Luca. Io credo che farà tante cose interessanti per la politica nazionale, ma questo che c'entra con la questione di costituzionalità? Attendevo con impazienza l'intervento del collega Giorgis, a cui sono veramente legato da un sentimento di stima per la sua qualità giuridica. La mia domanda era: perché c'è la questione di costituzionalità? Perché allora domani sono pronto con un intervento sull'esercito russo in Italia, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi malfunzionanti, ma garantiti da un ex Presidente del Consiglio; sono pronto a parlare di questo domani. È un anticipo: domani parliamo di questo.

bisognerebbe che la Commissione d'inchiesta si allargasse alle Regioni, che è un tema che condivido. Se si fosse allargata alle Regioni, sarei stato contento. Quando si è votato in Lombardia, la maggioranza di centrodestra ha eletto presidente della Commissione d'inchiesta una di Italia Viva. Siccome la minoranza di centrosinistra non voleva un rappresentante di Italia Viva, ma voleva uno del centrosinistra, ho chiesto a quella di Italia Viva di dimettersi. Si è talmente dimessa che si è dimessa da Italia Viva. Il collega Alfieri sa bene di che cosa sto parlando. Siccome è andata così, non venite a raccontarci che c'è una questione di costituzionalità, perché non si parla della Lombardia. Della Regione Lombardia abbiamo discusso in Lombardia. Si poteva discutere anche qui. Certo che lo si poteva fare anche qui e si è scelto di non farlo. Questo è un *vulnus* della Costituzione? Allora andiamo sulla sentenza che avete citato tutti, perché le sentenze vanno lette tutte fino in fondo: la sentenza n. 231 del 1975. Tutti e tre avete citato la sentenza. Non è che hanno mancanza di fantasia, signor Presidente, ma semplicemente è la sentenza chiave: lì si dice giustamente che il compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è di giudicare e nessuno di noi vuole giudicare né Conte, né Speranza, né Fontana. Nessuno. quello di raccogliere notizie: l'avete citato tutti e tre nello stesso modo e francamente sembrava che vi foste messi d'accordo. Tutti e tre vi siete però fermati su un punto: «per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso» e vi siete fermati lì. Io ho avuto la fortuna di leggere la frase di questa sentenza - le sentenze vanno lette tutte, specie quelle della Corte costituzionale - che dice: «L'attività d'inchiesta rientra, insomma, nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche». Onorevoli colleghi, noi abbiamo fatto 97 Commissioni di inchiesta e non facciamo una Commissione di inchiesta su un evento che ha visto la deroga di tutti i principi costituzionali? Penso che si sia fatto bene, e stavo in maggioranza in quel momento: si è derogato non a un articolo della Costituzione, tutti i principi costituzionali sulla libertà in nome di un principio di salvezza nazionale e di sanità. Tutto legittimo. Ma, se a fronte di questo, a fronte di appalti in deroga fatti da un'autorità commissariale che ha comprato per miliardi, non si fa una Commissione di inchiesta, come sulle modalità con le quali si sono chiuse le scuole (giusto o non giusto, non entro nel merito); se a fronte di un evento che ha portato migliaia di ha prodotto una chiusura del Paese e ha profondamente lacerato il sistema del nostro Paese - non per fare un giudizio penale nei confronti dei Ministri, perché nessuno di noi ha la minima intenzione di fare un giudizio penale - il Parlamento diserta il Parlamento diserta e non ha il coraggio di andare ad approfondire quello che è successo, non è che il Parlamento fa una scelta politica: il Parlamento fa una scelta di vigliaccheria istituzionale verso il futuro. *(Applausi)*. Vi dico che cosa penso io e chiudo: a me non interessa andare a rivangare quello che è successo sul passato. Io i conti col passato li ho fatti nel momento in cui, per la mia parte politica, ho lottato per un cambio di Governo e ho fatto politica. I conti con il futuro si fanno prendendo atto di quello che è successo e dicendo alle nuove generazioni: abbiamo fatto bene qui, ma abbiamo sbagliato qui e lì. Che paura può farvi la verità su questi fatti? E, soprattutto: qual è l'argomento giuridico costituzionale per porre una pregiudiziale di costituzionalità? Il fatto che non si faccia una Commissione sulla Lombardia? Io metto agli atti che avrei preferito che si studiasse anche la questione delle Regioni. Metto agli atti che non ho alcun problema a parlare di tutto, nemmeno dei vaccini. Siccome credo nella scienza, sono orgoglioso di aver fatto parte di un Governo che ha aumentato i vaccini obbligatori prima che ci fosse la pandemia (non dopo) e ha difeso i virologi quando non andava di moda farlo. Ma proprio per questo, siccome non ho paura della verità, credo che sia assurdo porre una questione pregiudiziale di costituzionalità. Penso che l'onestà intellettuale - che ella, onorevole Giorgis, ha richiamato - porti a dire che queste questioni pregiudiziali vanno respinte in modo fortissimo.

che a parere nostro muove dall'incombenza di dover chiarire alcuni aspetti di quel breve ma lungo periodo della storia italiana, un momento tragico e drammatico, che abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle o sulla pelle dei nostri amici e dei nostri parenti. È vero: è un breve periodo, perché la pandemia è piombata sulle nostre vite improvvisamente, nel gennaio 2020, e ci ha accompagnato fino all'inizio del conflitto russo-ucraino all'inizio del 2022. Ma quel tempo, nella mente di ogni italiano, è stato lunghissimo, anche perché ognuno di noi ha temuto il peggio per sé e per i propri cari, in quanto nessuno di noi conosceva il nemico che aveva di fronte, né a quei tempi lo conosceva la scienza. La dimostrazione sta nel fatto che i primi vaccini sono arrivati dopo circa un anno; tanto, probabilmente poco, perché a tempo di *record* si sono riusciti, attraverso la scienza e la ricerca, ad attivare vaccini che ci hanno accompagnato e aiutato con un piano che ha dato i frutti che ci aspettavamo e che ci ha fatto uscire dal tunnel. Siamo però consapevoli dell'imprevedibilità di ciò che è successo, perché ciò che è successo ha trovato impreparati non solo noi come Italia, ma tutti i Governi e tutte le nazioni. Però sarà necessario comprendere perché non ci fosse un piano pandemico nazionale allo scoppiare della pandemia; per quale ragione non ci fosse uno strumento di cui ogni Stato dovrebbe essere dotato. Bisogna poi chiarire quale sia stato il ruolo delle mascherine, delle tanto vituperate e ricercate mascherine, il loro utilizzo, quali fossero quelle efficaci e quali no. perché ad esempio molte scuole, altro luogo importante di contagio, siano state dotate di un tipo di mascherine che sono risultate assolutamente inutili e inefficaci; inefficaci; quale sia stata la gestione dei dispositivi di sicurezza, il loro acquisto - perché no? - e la distribuzione delle strutture pubbliche. Va detto che la maggior parte degli italiani ha seguito le indicazioni della sanità pubblica, visto che dietro le decisioni del Governo c'erano le informazioni dell'Istituto superiore di sanità. Ci sono stati quindi dei piani vaccinali seguiti da milioni di persone. Decine di migliaia di persone, però, sono morte. Il dolore per la loro scomparsa è ancora presente e sarebbe anche fondamentale stabilire un numero ufficiale o perlomeno attendibile. Quanti sono stati i morti per questa pandemia? Quanti invece sono morti in conseguenza di altre cause? Tutto questo inoltre ha fermato la nostra economia, soprattutto il turismo, un settore che muove una fetta importantissima del nostro prodotto interno lordo, che è crollato complessivamente del 9 per cento Ci sono stati migliaia di posti di lavoro persi, attività commerciali chiuse, attività economiche che hanno visto il proprio giro d'affari crollare. In conseguenza di un'economia di emergenza, si sono dovuti adottare decreti a sostegno delle attività economiche e a sostegno dei redditi dei cittadini, e li ricordiamo tutti. Va poi verificato quali siano stati gli effetti sulla rete sanitaria di prevenzione e di controllo delle altre patologie e quali siano stati gli effetti sulla salute dei cittadini italiani: liste di attesa saltate e controlli specialistici, per patologie anche gravi, non attuati nei tempi dovuti (lo ricordiamo tutti). La pandemia ha svelato quali fossero le debolezze e le fragilità del nostro sistema sanitario, sì. La crisi ha rivelato anche quali fossero i punti deboli del nostro sistema economico. Una valutazione serena in una Commissione parlamentare in cui siedano tutte le forze politiche va fatta e per diverse ragioni. La prima è quella di fare chiarezza e di fornire numeri precisi agli italiani che non siano manipolabili, ma che abbiano anche un crisma di certezza se non di scientificità. Ma la seconda è anche quella di capire se questa esperienza nefasta è servita o potrà servire a mettere assieme le competenze per affrontare meglio un'eventuale nuova pandemia, che chiaramente nessuno di noi si augura. Se non si danno certezze sui numeri, sui ruoli, sulla gestione di un evento tragico mai visto prima, non saremo in grado di affrontarlo con la dovuta preparazione qualora riapparisse. Voglio ricordare che Forza Italia in tutte le fasi della pandemia ha dimostrato grande senso di responsabilità, anche in quest'Aula, sia all'interno delle istituzioni che nel Paese, e ha rivelato un equilibrio nelle decisioni e nella comunicazione che, volto a far comprendere agli italiani la reale portata dei problemi da affrontare, non ha mai visto la nostra posizione politica fare passi indietro. Voglio infine rammentare che - lo ricordo agli amici dell'opposizione lo stesso Parlamento europeo ha istituito una Commissione d'inchiesta per analizzare i fatti e le conseguenze del Covid-19 e farne tesoro per un'eventuale pronta risposta delle istituzioni europee. I parlamentari di Forza Italia parteciperanno quindi con serietà e in modo responsabile ai lavori della nuova Commissione e sono decisi a dare il proprio contributo e le proprie idee. Per questo annuncio il voto contrario alle tre pregiudiziali presentate.

dalla minoranza, in quanto riteniamo non abbiano fondamento da un punto di vista tecnico e costituzionale, come messo in evidenza, e anche per delle ragioni naturalmente politiche. mio parere - puntare l'indice sul fatto che siano le Regioni le responsabili di tutto quanto accaduto, perché il Sistema sanitario è diverso delle Regioni in quanto la tutela della salute è una materia concorrente, così come previsto dal Titolo V della Costituzione. Perché dico questo? Prima di fare questa affermazione, che indubbiamente è strumentale, bisognerebbe capire

mise a capo della gestione dell'emergenza solo ed esclusivamente la figura del Presidente del Consiglio, con i famosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Quella norma, quel decreto, in nome di quell'emergenza, porta la gestione della pandemia in capo quindi, centralizza quella gestione. Voi citate indubbiamente il fatto che alcune Regioni abbiano preso delle strade diverse rispetto a quanto dava come indicazione lo Stato. tanto vero che poi la Presidenza del Consiglio faceva ricorso, si andava al TAR, nei tribunali, e la sentenza principe, che vi cito,

in buona sostanza è dello Stato il potere di gestione dell'emergenza sanitaria tramite l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ed è sempre dello Stato il potere di presidiare l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti. Quindi sostanzialmente la gestione della pandemia è stata centralizzata. Lasciamo perdere il discorso della sanità territoriale. Poi ognuno ha le sue responsabilità, perché anche a noi non interessa - e lo diciamo seriamente - puntare l'indice o processare. Ha detto bene il presidente Mattarella: non c'è un contropotere giudiziario del Parlamento, né tantomeno spetta al Parlamento valutare se una legge è conforme o meno alla Costituzione. A noi non interessa colpevolizzare, processare o puntare il dito al presidente Conte, al ministro Speranza, al Governo, anche perché quando si arriva ad affrontare uno *tsunami* di questo tipo chi può avere la verità in tasca? Chi può sapere come affrontarlo? Certo, si può prevenire, si può studiare, si può migliorare. Non lo metto in dubbio. Ma - attenzione - se processiamo la politica quando affronta le emergenze perché non lo ha fatto come sarebbe stato meglio, significa che un domani non troveremo più un politico che affronterà un'emergenza. Quindi, attenzione: noi non abbiamo nessuna intenzione di andare in questa direzione perché sarebbe controproducente.

quali sono stati gli errori che abbiamo commesso, tutti in buona fede, avendo votato dei provvedimenti in Parlamento, e cercare di evitare che non si ripetano in futuro. Perché la Corea e Singapore hanno affrontato in maniera più

proprio per far fronte a quelle che potevano essere ulteriori pandemie che potevano capitare o situazioni riguardanti la sanità. Questo è, resta e deve restare l'obiettivo non certo puntare l'indice e fare i processi. Ho ascoltato adesso le solite questioni e polemiche su Salvini che diceva "aprite tutto, chiudete tutto". Ricordo però che anche dall'altra parte sentivo dire che il virus non era contagioso, che bisognava andare nei ristoranti cinesi. Si misero a ridere quando il presidente il presidente Fontana indossò in mondo visione la mascherina, salvo dopo due settimane chiedere tutti perché non mettevamo le mascherine *(Applausi)*, gettando fango sulla Lombardia, sui camici bianchi, per poi dopo essere smentiti dalle sentenze, dai fatti e - signori - anche dai risultati elettorali. Faremmo prima tutti

e invece non ci si poteva assolutamente discostare da quello che era quel protocollo. Perché dopo un anno, non all'inizio, non si è appresa la capacità di tanti medici che avevano curato a casa i pazienti, avendo quel coraggio che a tanti è mancato, ottenendo anche dei buoni risultati evitando le ospedalizzazioni tanto quanto hanno fatto i vaccini, che hanno sicuramente avuto un ruolo importante e fondamentale per il superamento della pandemia e le forme gravi della malattia.

in tutto il pianeta, votandole, e nonostante questo non abbiamo avuto quei risultati sperati. Ci sono stati infatti Paesi che sono stati più morbidi e hanno ottenuto invece dei risultati migliori. Per quale motivo? Cerchiamo di capirlo senza dire che è colpa di questo o di quell'altro; alla fine abbiamo votato tutti - chi più, chi meno - i provvedimenti in quest'Aula. Magari io ne ho saltato qualcuno, perché su qualche questione avevo qualcosa da ridire, ma lo facevo sempre a titolo personale perché il mio partito ha sempre partecipato alle scelte nel bene

migliora, ma non è la verità assoluta, così come ci è stato imposto; a un certo punto era una religione, era una dea: era diventata la dea che faceva i miracoli. Allora vogliamo cercare vogliamo cercare di capire tutto questo per evitare che un domani si possa ulteriormente ripetere e per migliorare il nostro approccio, sicuramente scientifico, sicuramente di comunicazione, sicuramente legislativo, sicuramente burocratico, perché c'è stata anche la burocrazia del Covid e a un certo punto c'era una norma che contraddiceva l'altra. Possiamo fare questo? Penso che il compito del Parlamento vada proprio in questa direzione: con calma, serenità e trasparenza cercare di capire gli errori, così la prossima volta saremo - noi o chi verrà dopo di noi - nelle condizioni di poter fare decisamente meglio, aiutando la nostra popolazione. Signor Presidente, già il collega Giorgis ha espresso bene le ragioni per le quali noi voteremo a favore della pregiudiziale Ricordo che la pregiudiziale riguarda non solo ragioni di illegittimità costituzionale presunta di provvedimenti, ma anche ragioni di merito, quando si ritengono ragioni così forti da consigliare di non esaminare i provvedimenti. Questo lo dico perché ho sentito parlare prima di questioni di sola legittimità costituzionale. Certamente una Commissione di inchiesta che analizzi i fatti che hanno accompagnato la gestione di un evento così drammatico e inedito nella storia non solo italiana ma del mondo, come la pandemia da Covid-19, potrebbe essere una scelta corretta e oculata. tratta infatti di un episodio che ha segnato indubitabilmente le nostre vite e ha messo anche a nudo tante difficoltà, e non solo del nostro Paese, ma di tutti i servizi sanitari del mondo nel fare i conti con un virus imprevedibile e imprevisto. Tuttavia, le ragioni per le quali noi riteniamo che non si possa procedere con questa Commissione così come elaborata sono state sono state spiegate con chiarezza dal collega Giorgis e anche dagli altri intervenuti prima di me. Non si può fare una Commissione, che avrebbe il compito di verificare i fatti, di analizzare i dati, di comprendere cosa è successo, senza consentirle di poter esaminare tutto

sia tutto quello che è stato fatto a livello regionale. Non è solo una questione di polemica politica, perché il Governo era di un certo colore e le Regioni era di un altro colore. Il problema è che le Regioni avevano e hanno una competenza decisiva sul tema della sanità e l'hanno avuta anche nel momento della gestione della pandemia. Lo sappiamo tutti: le Regioni hanno

delle funzioni che le sono assegnate dalla Costituzione. Se non consentiamo alla Commissione di esaminare con chiarezza tutto quanto è accaduto, comprese le gestioni delle singole Regioni, non le consentiamo di fare un lavoro accurato.

che questa Commissione serva solo come strumento di battaglia politica e non è ciò che serve al Paese. Desidero fare un esempio molto chiaro della ragione per la quale

il 28 febbraio a Brescia c'erano 57 ricoverati in terapia intensiva; il 9 marzo, nove giorni dopo, i ricoverati in terapia intensiva erano 440. In quel momento a Brescia e in tutta la Lombardia eravamo sott'acqua;

accanto a Brescia, nella Regione Veneto, in quel momento non c'era quell'emergenza, c'erano tanti posti letto disponibili: pensate che a metà marzo 2020 in Lombardia c'erano 700 ricoverati in terapia intensiva, in Veneto 50. C'erano tanti posti letto disponibili, eppure non ha funzionato la solidarietà interregionale.

Io non sto accusando nessuno, non voglio fare polemica politica, ne sto solo parlando di una circostanza che dovrebbe suggerirci di fare un'inchiesta vera, che ci faccia capire perché e cosa non ha funzionato anche a livello regionale, anche nella solidarietà mancata tra Regioni. Son queste le ragioni per cui riteniamo del tutto inutile e controproducente una Commissione d'inchiesta che servirà solo alla polemica politica e non ad aiutarci a ricostruire quanto è successo. È una Commissione d'inchiesta che serve a quello scopo e non al Paese.

onorevoli colleghi, prendo la parola perché oggi nei lavori del Consiglio comunale di Torino, la mia città, si è verificato un fatto che reputo grave grave per la storia del nostro Paese e di questo Parlamento, nel quale attualmente tutti sediamo e che cerchiamo di onorare. Cosa è successo? Oggi la Commissione toponomastica della mia città ha bocciato la proposta di intitolare un viale pedonale alla persona di Nilde Iotti. Credo che non occorra ricordare cosa è stata Nilde Iotti per il nostro Paese: ha rappresentato i livelli più alti delle istituzioni ed è stata parte fondante della storia della nostra Repubblica. *(Applausi)*.Di quale storia? Non solo di quella importantissima della scrittura della Costituzione - è stata una Madre costituente Madre costituente - ma è stata protagonista della scrittura della storia costituzionale della nostra Repubblica negli anni che vennero, della costruzione della nostra storia repubblicana, della nostra democrazia, della storia delle nostre libertà, del ruolo del Parlamento. Ha interpretato con imparzialità politica tutti i ruoli istituzionali che ha ricoperto. È stata la prima donna Presidente della Camera dei deputati; Presidente della Commissione bicamerale; Vice Presidente del Consiglio d'Europa; una figura di grande equilibrio e autorevolezza, alla quale noi oggi dovremmo tutte e tutti guardare.

femminile. Voglio dire che la storia di emancipazione che parte dalle donne, ma che ovviamente noi vogliamo che sia una storia di emancipazione di donne e di uomini, è il modo principale in cui si deve parlare di popolo. Quando si parte dall'emancipazione, il popolo diventa cittadinanza e questa è la nostra Costituzione. La figura di Nilde Iotti è stata un simbolo della storia patria, della storia patriottica in questo senso e lo voglio ricordare. Sono sicura che la figura di Nilde Iotti non rappresenti e non possa rappresentare un motivo di imbarazzo per i partiti della destra che oggi non hanno votato in Consiglio comunale l'intitolazione della strada a Nilde Iotti. *(Applausi)*. Ne sono sicura, perché tra l'altro vorrei ricordare a questa Assemblea l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha citato Nilde Iotti nel discorso del suo insediamento. E, quindi, sono sicura

per porre rimedio alla grave mancanza che si è verificata, che fa torto alla nostra storia repubblicana e alla storia della mia città, Torino, che è stata la prima Capitale d'Italia e città medaglia d'oro della Resistenza. *(Applausi)*.

desidero ricordare in quest'Aula i ragazzi di Trieste. Settant'anni fa, in questi giorni, le strade di Trieste, la mia città, si coloravano di sangue per una rivolta che nasceva nel nome del Tricolore. Trieste in quegli anni era una città contesa. Mentre l'Italia cominciava a ricostruirsi dopo la guerra, Trieste viveva la condizione angosciosa di città rivendicata. Dall'altra parte c'era Tito, c'era la Jugoslavia comunista che reclamava Trieste e aveva lasciato a Trieste il ricordo di un'occupazione, seguita a quella nazista, che aveva riempito le foibe del nostro Carso, che parlava di 4.000 scomparsi chissà dove. E aveva lasciato il ricordo tragico di quella quarantena, di quei quarantadue giorni in cui Trieste era stata dichiarata annessa alla Repubblica federale di Jugoslavia, in cui l'ora era stata adeguata all'ora di Mosca in cui, per l'appunto, si voleva portare via all'Italia quella Trieste sacra agli italiani. La rivolta di ragazzi di Trieste nacque non a caso, in un giorno sacro alla Patria. Il 4 novembre i triestini, gli italiani di Trieste, si recarono a Redipuglia in massa e di ritorno da Redipuglia tornarono nella città in cui li aspettava il generale inglese Winterston. La città era stata infatti confinata in un assurdo territorio libero voluto dall'infame Trattato di pace del 1947, che aveva diviso il cosiddetto territorio libero di Trieste in zona A, cioè la città di Trieste e quella che è oggi la sua misera provincia, e una zona B, che è la parte nordoccidentale dell'Istria, che era invece amministrata dalla Jugoslavia comunista. Ebbene, quei ragazzi tornarono e il generale inglese Winterton aveva proibito l'esposizione del Tricolore. I ragazzi tornarono sventolando la bandiera e tutto nacque lì. Un ufficiale inglese strappò la bandiera di mano ad un ragazzo e una ragazza, la più coraggiosa di tutte, si lanciò a testa bassa verso quel colonnello Da lì nacquero gli scontri del 4 novembre e furono scontri durati tutto il pomeriggio fino alla serata del 4 novembre. novembre. La mattina seguente le scuole di Trieste proclamarono lo sciopero e tutti i ragazzi uscirono dalle scuole e riempirono la città di bandiere Si svolgevano cortei spontanei ovunque e si ripetevano scontri sulle strade di Trieste, scontri continui. C'era il famigerato nucleo mobile della cosiddetta polizia civile, furono rovesciate camionette; questo accadde anche dopo e ci furono altri scontri violenti. I ragazzi si rifugiarono dentro la chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Questo accadeva al mattino. Gli inglesi spalancarono le porte del tempio, usando gli idranti, fecero entrare il nucleo mobile che, con i manganelli, riempirono di sangue la chiesa. Il vescovo di Trieste ordinò la riconsacrazione della chiesa. Era il pomeriggio del 5 novembre 1953. Quando i ragazzi e la gente di Trieste avevano riempito il tempio, arrivarono improvvisamente le camionette inglesi che circondarono

Pierino Addobbati. Era un ragazzo esule da Zara. Suo padre

Pierino Addobbati morì per primo. Ho incontrato qualche giorno fa suo fratello che vive ancora, mi ha abbracciato e mi ha detto di ricordare ancora quel giorno in cui fu la sua stessa mamma a mettergli la coccarda tricolore sul petto. Fu colpito proprio sul petto: lo colpirono all'aorta, aveva quattrodici anni e morì davanti alle scale di Sant'Antonio Nuovo. Ci sono ancora i buchi dei proiettili. Poco più in là moriva anche Antonio Zavadin, che era un marittimo di La notte fu drammatica e terribile; la mattina gli scontri ricominciarono. Gli inglesi fecero togliere anche il tricolore che aveva esposto il sindaco di Trieste, quello che diventerà poi il sindaco della seconda redenzione. Gli scontri si spostarono in piazza Unità, che era il luogo sacro di Trieste. Il primo a morire fu Nardino Manzi *(Applausi)*: quindici anni ed era esule da Fiume. Era il più coraggioso: in tutte le foto di quel giorno lo si vede avanzare per primo, con a fianco un altro coraggiosissimo, che si chiamava Francesco Paglia, aveva ventiquattro anni ed era il capo della Goliardia nazionale di Trieste. Vedete com'è la sorte: morì in piazza Unità, sotto la prefettura, strappando la carabina a un inglese, colpito da un cecchino dall'alto. Poco più in là, dall'altra parte della piazza, moriva Saverio Montano, un padre di famiglia di Ma la storia incredibile dei due è che Francesco Paglia era stato un bersagliere volontario nella Repubblica Sociale Italiana e aveva difeso il confine sulla Selva di Tarnova, sopra Gorizia. Dall'altra parte, Saverio Montano era un partigiano, ma era un partigiano bianco, non di quelli che volevano dare Trieste a Tito era un partigiano volontario della libertà. *(Applausi)*. Morirono insieme un fascista e un partigiano per Trieste italiana. E poi morì ancora Erminio Bassa, un barese. In quei due giorni morirono questi sei uomini e ragazzi che, per la mia generazione, sono stati un faro di eroismo, di bellezza, di splendore, di italianità.

Trieste tornava all'Italia e l'Italia tornava a Trieste. *(Applausi)*. Sono stati per noi gli ultimi martiri del nostro Risorgimento. Gli eroi non muoiono mai. Per me, per noi, il fatto di ricordarli ancora una volta settant'anni dopo, in questo Parlamento, è ricordare la bellezza dell'eroismo, la nobiltà della vita, la casa, l'amore, la patria, l'amore per la nostra adorabile Italia.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

causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2",

- Disegno di legge n. 825 - Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi